Onorevoli colleghi, nella giornata di ieri, nei pressi dell'aeroporto di Pisa, un aereo da trasporto dell'Aeronautica militare è precipitato nel corso di una missione di addestramento, causando la morte dell'intero equipaggio, composto da tre ufficiali piloti e due sottufficiali. La tragedia della morte prematura ed improvvisa di cinque nostri militari, nell'adempimento del loro dovere, ci rattrista profondamente. La Presidenza del Senato ha già avuto modo di rappresentare ieri, in un messaggio che è stato inviato al Capo di Stato maggiore dell'Aeronautica, generale Daniele Tei, i sentimenti del nostro comune dolore. La 46ª Brigata aerea, della quale facevano parte i cinque militari caduti, si è distinta in molteplici occasioni nello svolgimento di delicate missioni a carattere umanitario, nel campo dei soccorsi medici e della cooperazione sanitaria. Sono certo di interpretare i sentimenti di tutta l'Assemblea nel manifestare alle Forze armate, all'Arma dell'Aeronautica e, prima di tutto, ai familiari, il più vivo cordoglio e una sincera partecipazione al loro lutto, unitamente al caloroso e grato apprezzamento per l'operato, in Italia e all'estero, di tutti i nostri militari. *(Generali applausi).* Invito pertanto i colleghi ad osservare un minuto di raccoglimento.

Signor Presidente, mi associo, a nome del Partito Democratico, al cordoglio espresso dalla Presidenza del Senato

La nostra Aeronautica ha avuto negli anni passati momenti di difficoltà, con numerosi incidenti. Da molti anni si viveva invece un periodo più tranquillo; purtroppo più recentemente - già l'anno scorso e poi quest'anno - ci sono stati due gravissimi incidenti. Credo che, per il lavoro che dobbiamo svolgere in Commissione, dobbiamo seguire con estrema attenzione e con il massimo rigore il lavoro delle nostre Forze armate.

lo sforzo a cui sono tenuti tutti i nostri militari e la nostra presenza in ambito ONU, NATO e nelle missioni umanitarie in corso in tante parti del mondo, che ha fatto sì che tanti ragazzi lasciassero

alle famiglie, ai piccoli figli che i nostri militari lasciano e a tutti i compagni delle Forze armate - dell'Esercito, della Marina e dell'Aviazione che sono chiamati a compiere questi sforzi. Ad essi le istituzioni e il Parlamento devono far sentire la loro vicinanza*. *(PdL)*. Signor Presidente, il Gruppo del Popolo della Libertà, congiuntamente anche agli altri colleghi,

perché si vedono davanti a noi, si traguardano scenari di vite messe a disposizione della comunità nazionale

vivono e sentono il peso del particolare lavoro che svolgono i loro congiunti nelle continue attività di addestramento, nelle tante azioni condotte per la pace nel mondo

anche il Gruppo dell'Italia dei Valori si associa al dolore che ha colpito l'Aeronautica militare e le Forze armate per quanto accaduto ieri. Noi le siamo grati, signor Presidente, perché ha voluto ricordare la vicinanza del Senato alle vittime del dovere.

delega al Governo in materia di lavori usuranti, riorganizzazione di enti, congedi, aspettative e permessi, nonché misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico, di controversie di lavoro e di ammortizzatori sociali,

*relatore*. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, certamente non si può dire che il tempo che ha consentito a questo provvedimento, finalmente, di approdare in Aula sia stato breve,

grazie alla collaborazione dei colleghi della minoranza nelle Commissioni 1a e 11a, di svolgere un buon lavoro. Oggi noi sottoponiamo all'Assemblea un provvedimento la cui capacità d'incisione sulla grande crisi che ha alluvionalmente colpito il nostro Paese a partire dall'estate scorsa può essere davvero importante. Dei diversi provvedimenti che sono stati trasferiti da questa sua sede iniziale, determinando

la quale non è del tutto tradizionale rispetto all'impianto culturale del nostro Paese, perché cerca di allineare la strumentazione giudiziaria in materia di lavoro ai migliori standard internazionali. Il *focus* nuovo infatti è sulla conciliazione e sull'arbitrato intesi come strumenti per la valorizzazione del ruolo e dell'autonomia delle parti contrattuali e delle parti sociali. Questo è un *driver* che troviamo costantemente lungo tutto l'itinerario del provvedimento. ci sono passaggi forti per la tradizione italiana, perché valorizzazione dell'arbitrato significa valorizzazione dell'arbitrato anche secondo equità, e non soltanto secondo diritto; significa valorizzazione dell'arbitrato anche quando esso sia generato direttamente dal contratto individuale, anche se viene ovviamente realizzata una finestra di garanzia che consenta alle parti, con loro accordi, di intervenire per una regolazione che meglio indirizzi l'attivazione di tale strumento. È certamente nel senso della valorizzazione dell'autonomia delle parti contrattuali e sociali la norma che assicura la insindacabilità delle valutazioni tecniche, organizzative e produttive poste a sostegno di una decisione organizzativa dell'azienda in materia di attivazione del rapporto di lavoro, della sua risoluzione e della sua gestione, come durante i trasferimenti. Anche questo significa in qualche modo fermare una deriva antisindacale che tante volte era stata adottata dalla magistratura del lavoro, sempre intrusivamente sospettosa nei confronti delle determinazioni delle parti.

Si badi bene: non è una norma che si limita a ripristinare il vecchio assetto della legge Biagi; è che in questo momento è cruciale per le piccole imprese morsicate dalla crisi avere a disposizione uno strumento, come lo *staff leasing,* che consente alta qualità di prestazione professionale ed alta qualità di prestazione professionale strutturale, ma accessibile a basso costo per la configurazione organizzativa che lo *staff leasing* consente, mettendo a disposizione grandi e qualificati strumenti di gestione, senza dover pagare tutti i costi che il ricorso accidentale e congiunturale ad essi potrebbe determinare. Anche la materia previdenziale è stata oggetto di interventi di manutenzione propulsiva che alla fine rendono coerente il complessivo disegno

sincera, leale ed autentica affinché le parti possano rendersi ancor meglio protagoniste di una fuoriuscita dalla crisi che consenta al nostro Paese di tornare nell'aristocrazia industriale mondiale, un posto che gli compete e che potrebbe essere uno fra i risultati più inattesi, ma più densi di significato di questa brutta stagione.

L'Atto Senato n. 1167, infatti, si caratterizza per alcuni interventi normativi particolarmente incisivi in materia di rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione sotto certi aspetti, va a corroborare leggi precedenti, quali la riforma approvata con la legge n. 15 del 2009 e il successivo decreto legislativo attuativo. Gli interventi operati nelle varie branche della pubblica amministrazione riguardano la materia del diritto allo studio,

Più analiticamente, possiamo sostenere l'importanza dell'intervento in materia di diritto allo studio universitario: dall'entrata in vigore della Costituzione del 1948, si dà attuazione al diritto allo studio e all'accesso all'istruzione superiore con una delega legislativa attribuita al Governo, attraverso cui si individua un percorso di sostegno al diritto allo studio. Ed enfaticamente nella legge delega si ripercorre un po' la storia degli articoli 3, 33 e 34 della nostra Costituzione, in particolare del principio di uguaglianza materiale

eliminati gli ostacoli di ordine economico e finanziario che rendono il principio di uguaglianza non attuale.

prevedendo, per esempio, che anche i professori di seconda fascia possano godere dell'elettorato passivo per le elezioni di questi organismi. Un intervento ulteriore viene fatto sulla recente legge che ha ridisciplinato la materia concernente i ricercatori universitari. Parimenti vi è un ulteriore intervento in materia di mobilità del personale pubblico, prevedendo in particolare che, nei casi di trasferimento delle funzioni statali alle Regioni di trasferimento delle funzioni statali alle Regioni o agli enti pubblici, l'eventuale eccedenza dei pubblici dipendenti sia disciplinata dall'articolo 33 del decreto legislativo n. 165 del 2001,

i dirigenti (che rappresentano il datore di lavoro pubblico) devono informare le organizzazioni sindacali e queste possono chiedere l'esame del provvedimento, all'esito del quale poi i trasferimenti sono disposti sulla base di un criterio di mobilità ad istanza.

con l'articolo 8-*bis*, si affronta un tema particolarmente sentito dalle riforme precedenti in materia di pubblica amministrazione. della norma che corrobora la previsione già contenuta nella legge n. 15 del 2009 relativa alla totale trasparenza dei dati relativi ai dirigenti della pubblica amministrazione, tema particolarmente caro anche all'opposizione, in particolare al senatore Ichino, confermando in specie il principio di *total disclosure* previsto già da ordinamenti stranieri, quali quelli del Regno Unito, della Svezia, della Norvegia e dell'Europa continentale.

L'intervento è volto inoltre a tutelare la riservatezza relativa alle patologie dei pubblici dipendenti, prevedendo che, in caso di produzione di certificazione medica, debba essere sottaciuta solamente la diagnosi. Su questo punto credo che il provvedimento in esame sia molto importante e significativo e segni la differenza storica tra una visione della pubblica amministrazione organizzata sulla segretezza dei propri atti e sulla non trasparenza delle prestazioni dei suoi dirigenti per approdare ad un sistema totalmente pubblico e totalmente trasparente. trasparente. Signor Presidente, onorevoli colleghi, a questo risultato approdiamo tramite una norma legislativa, ma certamente le pubbliche amministrazioni avranno la possibilità di realizzare l'informazione più capillare

quello strumento fondamentale ed importante che è la partecipazione dei cittadini alla critica e alla giusta struttura della pubblica amministrazione. recenti tendenze, infatti, il tesoro nascosto delle società democratiche è costituito appunto dalla possibilità dei cittadini di partecipare all'organizzazione e al miglioramento dell'efficienza della pubblica amministrazione,

L'articolo 10 interviene sul conferimento di incarichi e l'attribuzione di funzioni dirigenziali, il successivo articolo 13 prevede una norma molto importante in ordine alla possibilità per i pubblici dipendenti di chiedere un anno di aspettativa per avviare attività professionali e imprenditoriali. In tale caso considerato agli stessi non si applicano le norme in tema di incompatibilità tra la funzione istituzionale e l'attività privata. L'articolo 14 corona il percorso straordinariamente importante e significativo di una rivendicazione avanzata dal comparto delle forze di polizia e delle Forze armate.

oggi non è stato normato sulla base delle riforme che hanno portato alla privatizzazione del rapporto di pubblico impiego. Ebbene, con il riconoscimento della cosiddetta specificità normativa si attribuisce al personale di tale comparto la possibilità di avviare politiche contrattuali e negoziali, ma soprattutto politiche di modifica legislativa degli ordinamenti ordinamenti idonee a perseguire una sostanziale equiparazione con il cosiddetto personale pubblico delegificato. Molto spesso in quest'Aula del Parlamento abbiamo ascoltato interventi diretti a sostenere le esigenze del personale di tale comparto; tuttavia, in questi interventi non è mai stata sottolineata l'urgenza di una norma di questa natura, conseguire l'obiettivo di equiparare, anche sul piano economico, normativo e funzionale, il personale statale in regime di diritto pubblico e il personale statale in regime non delegificato. Mi permetto di aggiungere, sull'articolo 14, relativo alla previsione della norma sulla specificità delle Forze armate che ulteriori provvedimenti normativi, in particolare finanziari, dovranno evidentemente rinvenire risorse aggiuntive che serviranno a remunerare questa attribuzione di specificità alle Forze armate e di polizia. Non è un caso che questa rivendicazione fosse dallo scrivente in una piattaforma rivendicativa circa vent'anni fa ed è una pura coincidenza che da parlamentare sia io stesso il relatore di tale importante conquista per il mondo delle forze dell'ordine e delle forze di polizia. L'articolo 17 interviene in materia di riordino dei congedi, delle aspettative e dei permessi e anche sulla rivisitazione e sull'individuazione di criteri oggettivi e soggettivi per l'attribuzione dei permessi relativi alla legge n. 104 nonché in materia di misure dirette a garantire l'esercizio di diritti a rilevanza costituzionale. L'articolo 18 modifica la legge n. 104 del 1992 in materia di portatori di handicap e interviene anche in materia di misure relative al sostegno della paternità e della maternità. Con l'articolo 19, di cui ho già detto, si prevede che il certificato di malattia debba contenere semplicemente l'attestazione della prognosi e non della diagnosi, a garanzia della tutela della riservatezza; si prevede inoltre anche per la pubblica amministrazione l'invio telematico da parte dei medici direttamente all'INPS. L'articolo 21, infine, interviene in materia di incarichi del personale del comparto sicurezza nella pubblica amministrazione, prevedendo per la prima volta

22-*bis* interviene in materia di requisiti di accesso ai gruppi sportivi delle Forze armate e delle forze dell'ordine. Si prevede per tutti la possibilità di accedervi al compimento dei 17 anni; si prevede inoltre, prima del compimento della maggiore età,

22-*ter* interviene in materia di ruoli tecnici della Polizia di Stato. Una norma di semplificazione permetterà al personale dei ruoli tecnici, che sono suddivisi sulla base dei settori di specializzazione, di concorrere anche a settori di non diretta e specifica specializzazione, rendendo l'intero settore tecnico-scientifico più plasmabile alle esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e, in particolare, di efficienza

di minoranza. Mi rivolgo a lei e ai colleghi, signor Presidente, per svolgere alcune considerazioni in rapporto a quelle svolte dal relatore Castro, il quale opportunamente ricordava che questo disegno di legge nasce da un progetto estremamente ambizioso presentato dalla maggioranza all'avvio della sessione di bilancio dello scorso anno. Tale progetto definiva il pacchetto sostanziale delle riforme con cui questo Governo si presentava all'appuntamento dell'innovazione del Paese; esso è rimasto sostanziale anche dopo lo stralcio di molte norme avvenuto materie sostanziali l'esercizio della delega sui lavori usuranti, il lavoro sommerso, le controversie di lavoro, la delega sugli ammortizzatori sociali, oltre a tutte le norme in materia di lavoro pubblico. Di quell'ampia ambizione riformatrice però, secondo noi, dopo oltre quindici mesi dall'avvio del dibattimento alla Camera e dopo un anno di trattazione da parte delle Commissioni riunite, resta molto poco. Di questo non possiamo che rammaricarci. Le questioni che attengono al lavoro, agli strumenti di tutela e valorizzazione del lavoro, alla promozione delle politiche di innovazione del mercato del lavoro e alla lotta al lavoro nero sono temi cruciali per garantire al nostro Paese una direzione di uscita dalla crisi economica, evitando che essa produca una crisi sociale altrettanto

contestualmente messo in evidenza alcuni dati gravemente negativi in materia di lavoro. Il nostro Paese vede una crescita della disoccupazione, in particolare della disoccupazione giovanile, che avanza molto più rapidamente rispetto agli altri Paesi e rispetto alla media OCSE. Il Paese è carente di un sistema di stabilizzatori automatici

per innovare il quale non bastano assolutamente, a nostro avviso, le misure inserite nel provvedimento, né la riforma o l'ampliamento delle competenze delle agenzie di somministrazione, né, tanto meno, la reintroduzione da sola dello *staff* *leasing*. Rispetto a questi temi cruciali per la ripresa economica e per il futuro del Paese, il provvedimento è estremamente deludente: reitera, infatti, i tempi della delega per la riforma degli ammortizzatori e e degli strumenti di innovazione nel mercato del lavoro e per l'introduzione di nuovi strumenti dell'occupazione, dilazionandola nel tempo di oltre 24 mesi. Inoltre, riteniamo inaccettabile che la delega sui lavori usuranti, che ancora non è stata attuata ad una distanza così ampia dalla sua definizione, venga recata in questo provvedimento con un limite importantissimo che rende sostanzialmente inesigibile l'esercizio del diritto soggettivo di accesso alla quiescenza anticipata in caso di accertamento dei presupposti e dei requisiti per ottenere Ci sono molte altre materie che vengono affrontate con deleghe, a nostro avviso, troppo ampie: tra queste, il riordino degli enti vigilati dal Ministero del lavoro, che è in sé misura certamente per migliorare l'efficienza e l'efficacia della pubblica amministrazione, viene definito in termini assolutamente generici. Pur apprezzando che sia stata puntualizzata, su proposta del Gruppo del Partito Democratico, la salvaguardia del principio di autonomia di ricerca e di di autonomia funzionale di questi enti, ancora sussistono pesanti rischi in termini di autonomia dei diversi livelli di competenza istituzionale e di possibili ricadute negative con riguardo all'occupazione e alla qualificazione professionale del personale impiegato negli Troviamo censurabili, inoltre, gli interventi in materia di contrasto al lavoro sommerso e di variazione dell'orario di lavoro. Si agisce in questo campo alleggerendo le sanzioni e introducendo un principio Per contro, nessuno sconto - consentitemi la sottolineatura polemica - viene fatto in materia di esercizio

al diritto all'autotutela dei lavoratori. L'enfasi che viene data ai contratti individuali, alla possibilità di certificare i medesimi e di appoggiare le procedure arbitrali, gestite per equità anche sui contratti individuali, supera una tradizione consolidata di riferimento alla contrattazione collettiva in queste materie che, a nostro avviso, è presupposto di tutela indispensabile per un equilibrio tra le parti in causa. Su questo interverremo più dettagliatamente in sede emendativa. Concludo dicendo che siamo in un momento molto particolare, in cui tutto ciò che attiene al lavoro è di estrema delicatezza e determinante per il profilo con cui il Paese si presenterà all'uscita dalla crisi.

è un'altra cosa:

in questa direzione, ma non vi sono assolutamente investimenti in termini di risorse, come invece era stato fatto precedentemente. Pertanto, di per sé è soltanto una norma che invoca determinati criteri, ma che non produrrà risultati.

dall'amministrazione cambiando, in corso d'opera, non solo il diritto acquisito, ma anche tutto il percorso personale e familiare che si era deciso di compiere.

della necessaria cautela rispetto ad attività che il pubblico dipendente potrebbe svolgere una volta in aspettativa, magari anche in contrasto con gli interessi legittimi dell'amministrazione oppure utilizzando informazioni, posizioni

che dovrebbe provvedere alle pari opportunità, al *mobbing*, all'antidiscriminazione e al benessere dei lavoratori.

dei provvedimenti per l'alluvione in Piemonte. Addirittura, si istituisce la Commissione per la vigilanza e il controllo sul *doping* e per la tutela della salute nelle attività sportive.

i limiti minimo e massimo di età per il reclutamento degli atleti dei gruppi sportivi delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono fissati, rispettivamente, in diciassette Che cosa c'entra tutto ciò con un provvedimento che riguarda i lavori usuranti, la riorganizzazione di enti,

Un profilo di critica riguarda poi la circostanza che il provvedimento

si incide sull'attività parlamentare tipica dell'Aula,

necessitava di un tempo congruo per gli interventi emendativi.

Addirittura nell'articolo 28 si è intervenuti

l'intervento di una legge delega su una materia, il Parlamento di fatto viene privato della possibilità di intervenire in quella stessa materia. Ebbene, da oltre due anni anni non possiamo intervenire in materia di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione e apprendistato e di occupazione femminile, perché è materia di delega.

Così come è assolutamente incomprensibile il motivo per cui si interviene in materia processuale civile

mentre la Commissione giustizia esamina questa tematica, si interviene con un provvedimento e con norme estrapolate da un testo, spogliando la Commissione dei suoi dei suoi poteri ed affidandole quindi un ruolo solo consultivo. È chiaro che ci stiamo adagiando su due caratteristiche che contraddistinguono questa legislatura: l'eccesso della decretazione d'urgenza e l'uso abnorme della delega. Si tratta di intervento legislativo che snaturano, entrambi, il Parlamento. Quando si abusa della decretazione d'urgenza e quando vi è l'eccesso della normativa di delega, spesso in bianco, si espropria il Parlamento della sua funzione prioritaria, che è quella di fare le leggi. Il Parlamento

che cosa si vuole fare, nelle materie più strane e più complesse, saltandosi da un argomento all'altro. Questo non è un collegato alla finanziaria, è un'altra cosa: è l'ennesimo provvedimento *omnibus*, dove chiunque mette qualcosa. Ma in questo modo la nostra Costituzione è violata. Ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento,

tribuna una delegazione di studenti della Facoltà di Scienze politiche dell'Università di Genova. A loro rivolgiamo il saluto del Senato e gli auguri per la loro attività di studio. sulla questione pregiudiziale, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, potrà intervenire un rappresentante per Gruppo per non più di 10 minuti.

Signor Presidente, per il caso che qualche collega non sia compiutamente informato sulla materia su cui siamo chiamati a discutere e decidere, vorrei fare soltanto un rapido elenco degli oggetti di questo disegno di legge. Si parte dai lavori usuranti, per passare agli enti vigilati dal Ministero del lavoro, alle direzioni scientifiche degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, alle attività sportive, alla produzione di farmaci emoderivati,

*dulcis in fundo*, addirittura ad una norma di diritto processuale civile. Credo che sia la prima volta nella storia del nostro Parlamento che si propone e si porta a compimento una riforma del diritto processuale che non è passata per la sua sede naturale, cioè la Commissione giustizia.

cerca di farlo - noi stiamo creando un mostro legislativo, proprio il prototipo del provvedimento che non bisognerebbe emanare.

anche quelle cruciali e rilevantissime, come il diritto del lavoro ed il diritto processuale del lavoro, perché dobbiamo legiferare in questo modo? Farò solo due esempi di come questo modo di legiferare sbagliato nel metodo porti a risultati paradossali e assurdi nel contenuto: abbiamo appena varato la riforma delle amministrazioni pubbliche; adesso, a poche settimane di distanza, torniamo sulla materia dell'impiego pubblico. Abbiamo varato una riforma che mira a responsabilizzare la dirigenza pubblica rafforzandone le prerogative, ma qui all'articolo 9

nella legge n. 15 del marzo scorso e poi nel decreto delegato che ne è derivato. Sulla mobilità dei dipendenti pubblici interveniamo con l'articolo 8, stabilendo che un dipendente possa essere messo in mobilità quando rifiuti per due volte un trasferimento giustificato; nella riforma che abbiamo approvato nel marzo scorso, però, avevamo stabilito che le prerogative del dirigente su questo terreno dovessero essere le stesse che si applicano nell'azienda privata, dove basta un rifiuto ingiustificato perché scattino le sanzioni e il lavoratore debba rispondere del proprio rifiuto ingiustificato. Come la mettiamo? Che senso ha legiferare a singhiozzo come stiamo facendo? Il disordine consente che passino norme non coerenti con un disegno di riforma organica. Per questo ci sembra

un processo che necessita di tempi rapidi e che, quando fu introdotto, doveva essere celebrato all'insegna della celerità e della immediatezza. Questo provvedimento inoltre, che tende, a dare poteri consistenti e significativi

la necessità di un provvedimento più mirato, più preciso, più puntuale e minuzioso, che possa regolamentare fattispecie spesso difficili.

in materia di ammortizzatori sociali, siamo intervenuti a seconda delle necessità che la crisi imponeva e che vi è una necessità di inquadrare tutta la materia alla luce di un panorama finanziario ed economico globalizzato, che ha imposto nuove logiche, nuovi metodi e nuove strutture. Quindi, vi è la necessità di riguardare questo strumento,

il progetto di ammodernamento del Paese, disegnato con la finanziaria dello scorso anno, si va pian piano compiendo. Il mosaico che porterà l'Italia tutta, da Nord a Sud, a reggere il

a proposito di lavori usuranti e di riforma del processo del lavoro, sta producendo parte di questa importante azione riformatrice che è attesa da larga parte dei cittadini e del Paese.

disciplina delle attività di lavoro particolarmente faticose e pesanti. Anche gli esponenti dell'opposizione più responsabile hanno espresso un giudizio di astensione, e quindi non di opposizione, sul provvedimento oggi in discussione. Se da questi atteggiamenti si vuol trarre un significato politico, in un momento di particolare asprezza nel confronto tra le parti, esso è che non

una conquista per tutti. Credo che l'atto in discussione contenga numerosi altri elementi positivi come, per esempio, l'aver incentivato il ravvedimento operoso di quanti commettono violazioni, prevedendo una sanzione amministrativa più lieve per coloro che, dopo aver utilizzato lavoro irregolare, abbiano successivamente regolarizzato il lavoratore stesso. Il voto favorevole al provvedimento mi sembra giustificato anche per le nuove disposizioni volte a razionalizzare alcuni profili del processo del lavoro, processo che oggi non si svolge con la celerità necessaria a garantire la posizione giuridica sia del lavoratore, sia del datore di lavoro. Una riforma, quella del processo del lavoro, attesa da anni e che le norme in discussione in qualche misura anticipano visto che favoriscono conciliazioni e arbitrati o addirittura attuano la legge Biagi sulla certificazione dei contratti. Un'ultima osservazione a proposito della semplificazione normativa che con questa legge si introduce senza intaccare le tutele: a chi pensa che si sia voluto aggirare l'articolo 18 dei lavoratori voglio dire che non solo fa peccato ma sbaglia proprio! Il fatto è che la pletora di leggi sul lavoro sull'impresa prodotta negli anni dal Parlamento poteva essere sostenuta solo dalle grandi aziende. Ora la realtà è cambiata, e da parecchio tempo:

Ancora una volta, allora, si scopre che le gabbie ideologiche e le lenti deformanti di pregiudizi ben radicati per alcuni sono la vera grande difficoltà di un Paese che ha come sola risorsa una imprenditoria diffusa e una grande voglia di fare impresa.

al Governo in materia di lavori usuranti, riorganizzazione di enti, congedi, aspettative e permessi, nonché misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico, di controversie di lavoro e di ammortizzatori sociali, bisogna parlare principalmente

a fronte di un corpo docente universitario di 63.000 docenti. Poco più di due mesi fa (settembre 2009), l'Eurostat ha diffuso i dati i dati del rapporto su scienza, tecnologia e innovazione in Europa: nel 2007, i 27 Stati membri hanno investito complessivamente poco meno di 229 miliardi di euro, l'1,85 per cento del PIL europeo; la stessa quota del 2006, nonostante l'obiettivo contenuto nella Strategia di Lisbona (risalente al 2009) di arrivare al 3 per cento entro il 2010. Per fare un confronto, negli Stati Uniti si è speso il 2,67 per cento del PIL; e nel 2006, l'ultimo anno per cui ci sono dati disponibili, il Giappone ha speso il 3,40 per cento del PIL. In Europa solo due Paesi hanno rispettato gli impegni di Lisbona, raggiungendo e superando il 3

Fanalino di coda è Cipro, con lo 0,45 per cento. Guardando i valori assoluti, fa riflettere che tre nazioni da sole rappresentano il 60 per cento degli investimenti: si tratta della Germania con 62 miliardi, della Francia con 39 miliardi e della Gran Bretagna con 37 miliardi (l'1,79 per cento del PIL). Per l'Italia, dati riferiti al 2006 (non sono disponibili quelli relativi al 2007) indicano che la spesa era allora di 16,831 miliardi di euro, ossia l'1,13 per cento del PIL. Ma di che cosa parlate, signori della maggioranza? Questo è un Governo miope, che, oltre ad avere tagliato ulteriormente i fondi alla ricerca, tiene in vita, quasi ibernandole, le classi di potere e le baronie più vecchie d'Europa, aumentando ad esempio l'età pensionabile dei magistrati, che si vuole portare da 75 a 78 anni. Nel mondo universitario, nel dicembre del 2007, l'età media dei ricercatori era di 44,9 anni, quella dei professori associati di 52,1 anni e quella dei professori ordinari di 58,7 anni. Così, mentre orde di famelici baroni si godono il bel Paese, i giovani sono costretti ad emigrare per cercare lavoro, specialmente nel mondo accademico. Tale problema affligge in particolar modo la ricerca, dove i coraggiosi che provano a fare carriera in Italia sono ridotti a macchiette di anziane baronie. Ho voluto fare questa premessa per introdurre la questione dell'esercito dei precari, pari ad oltre 3,5 milioni, in gran parte lavoratori autonomi, ma anche dipendenti nei servizi pubblici, in maggioranza donne, ossia 58,7 e soprattutto meridionali, secondo l'ultima analisi della CGIA di Mestre (voglio ricordare che il ministro dell'economia Tremonti si fida più di loro che di altri istituti di ricerca più blasonati). Su un totale di 3.525.672 precari, è la Calabria, con il 23,3 per cento, a presentare il valore più alto, se viene preso come indicatore l'incidenza percentuale dei precari sul totale degli occupati presenti in ciascuna Regione.

Chiude la classifica la Lombardia, che, nonostante registri in termini assoluti il numero più elevato, presenta la percentuale più bassa sul totale degli occupati, ossia il

Chiude l'intermediazione finanziaria, con l'8,9 per cento. Infine, l'incidenza percentuale dei lavoratori precari per titolo di studio sul totale degli occupati vede i senza titolo toccare la percentuale del 20

Questi sono i dati del precariato in cifre, di quell'esercito di invisibili che invecchiano, spesso a spese di quegli ammortizzatori sociali che non date voi, signori del Governo, ma che sono rappresentati dalle famiglie, dagli anziani, dai vecchi che si devono fare carico, con le loro pensioni, di assicurare dignità ai giovani, a quell'esercito di precari. Sempre citando i dati,

provenienti da esperienze lavorative precarie terminate ed in cerca di nuova occupazione, per un totale di 3.757.000 lavoratori. Nel loro studio i ricercatori evidenziano anche che non sempre un periodo di lavoro flessibile diviene l'anticamera a forme contrattuali più stabili, ma che anzi con il passare del tempo dall'introduzione di queste forme lavorative «il tasso di conversione di occupazioni precarie verso lavori stabili è sempre più basso e il momento della trasformazione del contratto sempre più posticipato nel tempo» e che tra i precari non sono presenti solo giovani alle prime esperienze lavorative, ma vi è anche una non trascurabile presenza di *over* 40. La ricorrenza di tipologie di lavoro diverse dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato (lavoro a tempo determinato, lavoratori socialmente utili, contratti di lavoro interinale e di somministrazione, collaborazioni coordinate e continuative ed incarichi di studio, consulenza e ricerca) nel pubblico impiego era quantificabile in 103.349 contratti a tempo determinato, di formazione lavoro, 9.067 contratti di somministrazione e di manodopera e 34.457 lavoratori socialmente utili. Vi risparmio le altre percentuali.

Qui dentro ci sono disposizioni in tema di sanità (articoli 2-*bis* e seguenti), disposizioni in tema di università (articoli 6-*bis* e seguenti), disposizioni in tema di difesa (articoli 21 e 22-*ter*), arbitrato e conciliazione nel processo del lavoro modifiche al decreto legislativo n. 276 del 2003, la cosiddetta legge Biagi (articoli 28 e seguenti). Questa delega al Governo ha l'obiettivo di mettere mano alle pensioni dei lavoratori impegnati in attività definite usuranti, puntando a mettere in campo una vera e propria clausola di salvaguardia, che avrebbe lo scopo di evitare che troppe domande di pensionamento anticipato facciano sforare la copertura finanziaria a disposizione. Mi accingo alla conclusione perché il tempo sta scadendo. scadendo. Più che un diritto le norme sul lavoro usurante potrebbero diventare una lotteria. È già dura riuscire a rientrare nei parametri richiesti. Ad esempio, il lavoro notturno è considerato usurante se si fanno 80 turni notturni ogni anno; con il sistema degli orari basta un'influenza: si salta una notte e diventa in pratica impossibile arrivare alla quota richiesta.

il provvedimento che con alterne vicende giunge finalmente al nostro esame contiene importanti innovazioni per il mondo del lavoro sotto vari aspetti. Mi preme sottolineare innanzitutto le novità in materia di cause di lavoro, con l'introduzione della conciliazione davanti agli uffici provinciali del lavoro che, di fatto, semplificherà e velocizzerà notevolmente la soluzione delle controversie, con vantaggio evidente per i lavoratori, che potranno raggiungere un accordo e far valere le proprie ragioni senza dover perdere tempo e denaro nell'affrontare una causa. Al contempo sono state introdotte nuove e rilevanti disposizioni in materia di università, docenti e ricercatori, che prevedono la stabilizzazione dei pubblici dipendenti precari e hanno effetti anche sul personale tecnico‑amministrativo delle università. Atteso che dal 1° luglio prossimo le pubbliche amministrazioni non potranno più stipulare contratti a tempo determinato, è senz'altro positivo che le stesse amministrazioni dovranno trasmettere alla Presidenza del Consiglio l'elenco del personale in servizio assunto con contratto a tempo determinato, indicando la qualifica posseduta, la data d'inizio del rapporto di lavoro, nonché le eventuali proroghe e rinnovi, per consentire di monitorare costantemente la situazione. Si valuta positivamente, specialmente in un momento in cui è necessario ridurre le spese nel rispetto dei criteri di stabilità finanziaria, limitando un eccessivo ricorso - come in passato - al personale con contratto a tempo determinato, la possibilità di una riserva di posti (non superiore al 40 per cento) per i concorsi da bandire nel triennio 2009-2011, soprattutto al fine di valorizzare le esperienze e le competenze professionali acquisite. Un ulteriore aspetto positivo attiene alle disposizioni in materia sanitaria finalizzate ad assicurare l'indennizzo per complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie.

Riteniamo che nell'insieme queste norme comporteranno, da una parte, una semplificazione dei rapporti di lavoro tra le parti, dall'altra, una maggior tutela dei soggetti deboli. È per questo che ci auguriamo che finalmente,

durante l'esame in Commissione sono state eliminate dal testo una quantità di voci principali in tema di lavoro: gli articoli 3, 6, 7, 10, 15, 16 e 20 sono confluiti, su richiesta del ministro Brunetta, all'interno di altri provvedimenti, altri argomenti le norme sono state riformulate in modo diverso da come erano state concepite inizialmente. In questo non ci sarebbe nulla di male: l'attività parlamentare serve anche ad affrontare argomenti con una certa capacità di rimessa in discussione critica, per carità; sarebbe forse terribile se non ci fosse la capacità di capacità di addomesticare, secondo ragione, argomenti che richiedono di essere trasformati. Vorrei insistere soprattutto su uno o due temi che, al contrario, all'interno di questo *corpus* totalmente eterogeneo, mantengono un proprio punto di vista

neoliberista. Essenzialmente si tende a dare via libera alla logica dell'incontro, cosiddetto libero, nell'ambito del mercato, nell'ambito del mercato, e in questa maniera si sostiene che si aprano orizzonti di nuovi tipi di confronto nel sociale. Francamente,

il provvedimento mira a rafforzare e a valorizzare l'autonomia delle parti. Per carità, questa sorta di cammino, di passo indietro che lo Stato farebbe di fronte alle forze del mercato, forse, per certi aspetti, potrebbe essere considerato portatore di un profilo progressivo, ma mi chiedo questo rafforzamento e valorizzazione dell'autonomia delle parti faccia i conti con la diversità delle parti. parti. Immagino una piccolissima azienda produttiva dove il datore di lavoro e il lavoratore, come spesso accade in Italia (sono milioni le piccole aziende di questa natura), lavorano fianco a fianco,

si lasci campo libero al confronto autonomo delle forze. Tuttavia, se ciò si verifica su un terreno dove la bilancia delle forze è totalmente sperequata a favore dell'azienda,

abbiamo invece una situazione in cui l'azienda viene favorita proprio perché ha di fronte degli interlocutori deboli. Anzi, vorrei spingermi più in là.

il datore di lavoro, una forza collettiva e una forza singola. Io ritengo che l'analisi sociale degli ultimi decenni accrediti molto di più un ritratto completamente rovesciato: rovesciato: la condizione generale della precarietà del lavoro ha determinato una sorta di isolamento fisico, atomizzato, delle forze di lavoro. Il lavoratore spesso è solo nel mercato del lavoro: solo proprio fisicamente, non sostenuto nemmeno da forze collettive come il sindacato, o associazioni o protezioni volontaristiche di qualche tipo. Il lavoratore precario in modo

Che destino può avere una persona che sottoscrive un contratto in condizioni di estrema debolezza? Per spingermi ancora oltre, in in certe condizioni di lavoro universitario - ci ritorneremo perché purtroppo ne avremo l'occasione - si verifica addirittura una sorta di prerequisito che corrisponde alla sottoscrizione di un contratto di lavoro a titolo gratuito. Che cosa contratta una persona una volta che ha sottoscritto un contratto a titolo gratuito? In realtà, le forze lavoro non difese sono distribuite lungo un ampio campo di variabilità, a

a Roma direbbero come un sorcio - per poi sperare di riuscire a trovare in qualche forma una via. Questa non è una speranza statisticamente valida. valida. È una speranza che conta soltanto sulla capacità di autocostruire la propria fortuna da parte di pochissime persone. Gli altri sono gli abbandonati, gli indifesi, i solitari. che noi stiamo inconsapevolmente - o forse, ancora peggio, consapevolmente, da parte della maggioranza - costruendo una ginnastica delle libere forze del mercato in cui la libertà è tutta da una parte e la necessità tutta dall'altra, il caso tutto da una parte e la determinazione tutta dall'altra. C'è chi ha in mano la leva della dea Tyche e chi, invece, dipende dal destino altrui.

il provvedimento che giunge all'esame dell'Assemblea è un collegato alla manovra finanziaria per il 2009. Giunge, dunque, all'esame di quest'Aula con un notevole ritardo dovuto a continue interruzioni: basti pensare che la Camera dei deputati lo aveva approvato

o come le modifiche all'articolo 71 del decreto n. 112 del 2008, in materia di assenze per malattia dei pubblici dipendenti (exarticolo 20), anch'esse già in vigore con la legge Brunetta, o ancora come le disposizioni recanti proroghe degli ammortizzatori sociali (ex articolo 27) inserite nei cosiddetti provvedimenti anticrisi. sono state introdotte nuove rilevanti disposizioni, come quelle in materia di università, docenti, ricercatori, ovvero quelle in materia sanitaria.

una priorità nell'erogazione dei trattamenti qualora il numero delle domande accolte sia maggiore delle risorse finanziarie a disposizione; ciò a dimostrazione del fatto che questa maggioranza governativa è sensibile al tema dei lavori usuranti. al tema dei lavori usuranti. Sempre a tal riguardo, vorrei ricordare la battaglia condotta da parte della Lega per far rientrare all'interno dei lavori usuranti anche gli appartenenti alle forze dell'ordine, categoria che il legislatore deve considerare e tutelare, perché le forze dell'ordine garantiscono la sicurezza ai nostri cittadini. Per questo motivo, consideriamo l'articolo 14 del testo una vittoria, con particolare riguardo al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. Proseguendo nell'esame del provvedimento, per quanto concerne le cause di lavoro ritengo che le modifiche alle procedure di conciliazione siano importanti, perché facilitano sia i datori di lavoro sia, soprattutto, i lavoratori nel raggiungere un accordo evitando lunghe, estenuanti e costose cause.

una riorganizzazione della vigente normativa che, se non verrà strumentalizzata, porterà cambiamenti molto positivi per i nostri lavoratori e per i cittadini del nostro Paese. Per questo motivo, crediamo che esso debba essere portato avanti da quest'Aula senza ulteriori battute d'arresto. prima di entrare nel merito della discussione, che peraltro è durata oltre un anno, con improvvise fermate, riprese, salite e risalite,

anche questo è il segno di uno scarso rispetto nei confronti del Parlamento e di una grande confusione nel governare. Il provvedimento, collegato alla legge finanziaria per il 2009, arriva in quest'Aula, per quanto concerne questo ramo del Parlamento, dopo l'approvazione della legge finanziaria 2010: già questo dato dovrebbe dare la cifra dell'interesse del Governo verso tale provvedimento. Come in una sorta di scatola cinese, molte delle materie del disegno di legge sono apparse, poi scomparse, ed alcune improvvisamente ricomparse.

colleghi, i lavori usuranti sono una cosa importante perché si afferma il principio secondo il quale rispetto alla pensione non tutti i lavoratori sono uguali. Bisogna tenere conto per alcuni delle aspettative di vita - che per molti sono aumentate - ma per altri della gravosità, della fatica, del dramma e della pesantezza del lavoro fisico;

in strutture chimiche altamente inquinanti o in miniera, o con turni che investono il ciclo intero della giornata per una parte lunga e importante della propria vita lavorativa, e chi invece queste condizioni non le deve Così come si sta perdendo un'ulteriore occasione per definire, una volta per tutte, un sistema di ammortizzatori sociali degno di questo nome, in una situazione economica drammatica, con un tasso di disoccupazione crescente.

non se ne occupa; si occupa, invece, di impedire a due genitori, con un ragazzo diversamente abile molto grave, di poter usufruire di permessi contemporanei, come la legge prevedeva. prevedeva. Altre norme producono invece l'effetto di subissare di controlli inutili malati terminali. Questo è il rigore del ministro Brunetta, che non si occupa di consulenze e di altre disfunzioni, ma è rigorosissimo con chi ha *handicap* gravi e magari è un malato terminale. Ma il cuore di questo provvedimento riguarda le norme sulla conciliazione e l'arbitrato, che intervengono in maniera pesante sul ruolo della contrattazione e sul ruolo delle parti. In particolare, sull'arbitrato si passa dalla situazione attuale, di difficile applicazione, di fatto all'obbligatorietà dell'arbitrato stesso, con il rischio anche di violare precetti costituzionali sulla tutela giuridica dei diritti, come più volte ha affermato il collega Treu e come diranno meglio di me in sede di illustrazione degli emendamenti sia il collega Treu che il collega Ichino. Inoltre, voglio soffermarmi su un punto in particolare: cosa significa l'equità sull'arbitrato? Quando l'equità diviene parametro di giudizio? Cos'è l'equità? Come viene calcolata? A seconda del luogo? A seconda del giudizio? Quindi, quale uguaglianza di diritti per tutti i lavoratori?

che non hanno diritti; al lavoratore che è sempre più privo di tutele e con sempre meno garanzie. Si mette in discussione alla base il principio stesso di diritto individuale in tema di diritto del lavoro, mentre si attenuano le misure contro il lavoro nero e sommerso.

Per ultimo, volevo sottolineare le norme che sono apparse, scomparse e poi, a volte, riapparse. Le prime riguardano la lotta a chi usufruisce in maniera irregolare dei permessi o non fa il proprio dovere. Vorrei chiedere per l'ennesima volta al ministro Brunetta: quali sono i dati validi? Quelli che pubblica lui o quelli che pubblica la Ragioneria generale dello Stato? Forse l'irrequietezza e la perdita di *bon ton* che caratterizza le uscite di questi ultimi giorni del Ministro derivano dal fatto che dietro tutte le sue affermazioni, le sue grida, le sue continue interviste, nulla è cambiato. Semmai si sono accentuate la frustrazione e il distacco, sia dei lavoratori pubblici dal proprio lavoro, sia dei cittadini nei confronti dello Stato. Rispetto poi alle norme sulla stabilizzazione dei lavoratori precari, l'unica richiesta è questa: almeno non prendiamoli in giro. Così come non dovremmo prendere in giro il personale delle forze di polizia e delle Forze armate, cui continuiamo a togliere mezzi e risorse e non gli facciamo nemmeno i contratti! Ma questo è il tempo in cui il Governo vede il paese felice e tranquillo, come negli *spot* del "Mulino Bianco", mentre le condizioni delle persone sono sempre più drammatiche e si confrontano con la disoccupazione, la precarietà e i redditi bassi: centinaia di migliaia di lavoratori in cassa integrazione, che vivono con l'angoscia di non vederla rinnovata nei prossimi mesi e di non rientrare in azienda; centinaia di migliaia di lavoratori precari, che per primi sono stati esclusi dai cicli produttivi e che non hanno alcuna protezione sociale; i tanti precari della pubblica amministrazione e della scuola, che vivono con crescente angoscia il loro futuro occupazionale; milioni di nostri connazionali che vivono, o sopravvivono, sotto la soglia della povertà; povertà; le migliaia di piccole e medie imprese che rischiano di chiudere i battenti a causa della stretta creditizia in Italia e di una pubblica amministrazione che non funziona.

Signora Presidente, signori rappresentanti del Governo, onorevoli senatrici, onorevoli senatori, come bene i relatori hanno evidenziato, il disegno di legge arriva all'esame dell'Aula del Senato dopo un *iter* lungo e travagliato e presenta naturalmente al suo interno diversi tipi di intervento. Quando ho ritenuto di dover intervenire, ho fatto una valutazione su quale potesse essere il tema: o la generalità assoluta della necessità di una riforma complessiva man mano che questo Paese avanza, si evolve e, per quanto riguarda il contingente, supera la crisi; oppure cogliere, nell'ambito del disegno di legge, gli aspetti più significativi. Ritengo di dovermi soffermare su questi. Credo che il primo aspetto significativo di questo disegno di legge si abbia con l'articolo 8, relativo alla mobilità del personale delle amministrazioni pubbliche, là dove si dispone che, in caso di conferimento di funzioni statali

in vista dell'attuazione dell'ampio processo federalista, che questa legislatura ha avviato proprio partire dall'Aula del Senato, per cercare di evitare che, come spesso accaduto in passato, in occasione dell'attuazione di provvedimenti di decentramento amministrativo quale, ad esempio, la Bassanini, l'amministrazione statale non fosse di fatto nella condizione di trasferire, unitamente alle competenze funzioni, anche il personale necessario a svolgerle, con la conseguenza di determinare l'elefantiasi degli apparati pubblici, con personale oggettivamente sottoutilizzato ma confermato nei propri incarichi dall'amministrazione centrale, e personale da assumere *ex novo* nelle amministrazioni periferiche per svolgere le medesime funzioni.

nella sua relazione e riguardante il controllo giudiziale sul rispetto delle clausole generali contenute nella disciplina legislativa in materia di lavoro alla certificazione dei contratti di lavoro e alla valutazione da parte del giudice dei contenziosi concernenti i licenziamenti individuali). Considerate peraltro la rilevanza e in qualche misura la delicatezza del tema, ritengo più che comprensibile l'attenzione dedicata a questi passaggi della legge, anche con caratterizzazioni

all'accertamento del presupposto di legittimità e, nei commi successivi, con il rafforzamento vincolante anche nei confronti del giudice dell'accertamento effettuato in sede di certificazione dei contratti di lavoro.

nel valutare le motivazioni poste alla base del licenziamento, tenga conto, oltre che naturalmente delle fondamentali regole del vivere civile e dell'oggettivo interesse dell'organizzazione, anche delle tipizzazioni di giusta causa e di giustificato motivo presente nei contratti collettivi di lavoro, ovvero se stipulati dalle commissioni di certificazione nei contratti individuali di lavoro. penso che con quest'articolo e i successivi (il 24 e il 25) la norma intenda rafforzare il ruolo delle parti nella regolazione dei rapporti di lavoro, limitando nel contempo l'intervento del giudice del lavoro, che è chiamato a muoversi all'interno di precise indicazioni che scaturiscono dalla certificazione dei contratti. Si dà certezza: tali misure corrispondono all'esigenza, ma anche alla volontà di questa maggioranza, di rendere centrale nella controversia del lavoro il ruolo delle parti, dando valore cogente alle norme contrattuali liberamente stipulate, al fine di prevenire per quanto possibile il ricorso alle scelte giurisdizionali.

resta evidente nel nostro Paese la necessità di una riforma complessiva degli ammortizzatori sociali, che tenga conto anche dell'esperienza acquisita nella gestione dell'attuale crisi economica occupazionale, al fine di adeguare questi strumenti alla situazione attuale del mondo del lavoro. È una situazione che ha visto dilatarsi la tipologia dei contratti e l'emergere di nuove forme contrattuali, parallelamente alla crescita del comparto dei servizi, divenuto ormai decisamente più rilevante, per il peso occupazionale, di quello secondario (cioè di quello che fino a pochi anni fa era il sistema dell'industria). Quindi, agganciandoci, allo slogan: al lavoro per tutta la vita e non al posto di lavoro per tutta la vita (anche se con gli slogan si fa solo demagogia) , ritengo che questi temi, questi temi, caratterizzanti il disegno di legge, depongano a favore di una sua necessaria, tempestiva e definitiva approvazione, per dotare il Governo degli strumenti adeguati a una riforma complessiva di tutto il sistema degli ammortizzatori che, a mio avviso, dovrà caratterizzare in via prioritaria l'azione delle pubbliche istituzioni, non appena conclusa l'emergenza occupazionale indotta dalla crisi finanziaria mondiale, che ormai speriamo-

Signora Presidente, mi dispiace deludere ancora il collega ed amico Paolo Nerozzi, ma devo dirgli che sarò breve D'altra parte, trovo assolutamente singolare il principio, affermato dal collega Nerozzi, secondo il quale vi sarebbe una relazione diretta fra la serietà dell'analisi e la verbosità dell'analista. mi sembra un principio adatto a quei fumidi ed incupiti cineforum dove si trasmetteva, alla fine degli anni Sessanta, il film di Glauber Rocha «O' cangaceiro» che sono, probabilmente, uno dei luoghi del *Bildungsroman* dell'amico e collega Paolo Nerozzi ma che, francamente, mi sembrano poco adatti per il Parlamento. Lo dico, evidentemente, con tutto l'affetto che, invece, non ho trovato nel suo intervento, la cui acrità, francamente, mi ha sorpreso. Mi sembra che le argomentazioni svolte dagli illustri colleghi della minoranza si siano concentrate intorno ad un tema cruciale: se questo sia un provvedimento *omnibus* e, quindi se in qualche misura

questo è un provvedimento in collegamento con la finanziaria, il cui compito precipuo è quello di governare la grande crisi, possiamo noi sostenere che promuovere la certezza del diritto, concentrando il ruolo principale delle soluzioni delle controversie di lavoro nella conciliazione e nell'arbitrato non sia un rafforzamento di quella coesione sociale oggi decisiva per il superamento della crisi? Possiamo noi sostenere che limitare le incursioni giudiziarie dentro l'operato, dentro il perimetro liberamente presidiato dalle parti sociali, non sia un modo per rafforzare la loro capacità di innovazione e di governo attivo e propulsivo della crisi stessa? Come pensare oggi che le ispezioni, che accanto al momento meramente sanzionatorio vedono sottolineato anche il momento cooperativo e collaborativo, non siano anche esse uno strumento di rafforzamento di quella coesione sociale che oggi è vettore competitivo? La coesione sociale è un vettore competitivo, e questo è un provvedimento che alla coesione sociale guarda con grande certezza. Come dire, amici e colleghi, che razionalizzare 32 diversi tipi di aspettative e permessi non significhi condensare quella certezza del diritto che, a sua volta, è elemento propulsivo per una semplificazione che diventi agilità di gestione e possibilità, per la gestione stessa, di concentrarsi sulle aree più drammaticamente serie della risposta alla crisi? Proprio nel

il valore culturale delle produzioni, come non dire che, se vogliamo mantenere coesa la prospettiva del presidio dei costi, non possiamo non considerare salutare il ritorno dello *staff leasing*? Esso consente, infatti, anche alle piccole e medie imprese - lo ripeto - di avere competenze a prezzi che altrimenti non sarebbero per loro disponibili. allora, se questo è vero, credo che si tratti di un provvedimento sinceramente leale rispetto alla natura di una finanziaria che deve presidiare in modo articolato le prospettive della crisi. un'ultima osservazione nei confronti del collega Pardi, le cui considerazioni ascolto sempre con grande attenzione e curiosità intellettuale, perché spesso esse sono felicemente originali. invece dirle sommessamente, professore, che ho trovato una sorta di pregiudizio retorico nella sua argomentazione, come se in qualche misura il mondo fosse ancora diviso per classi gerarchicamente ordinate

che favorire l'invasività del giudizio ordinario - costringendo cioè il lavoratore, l'operaio della catena, della piccola impresa artigiana ad un processo che dura 12 anni sia più dispiegatamente democratico e attento alle ragioni del contraente presunto più debole, rispetto ad un arbitrato in cui, invece, le ragioni dell'operaio sono rappresentate dalla sua associazione sindacale, in un giudizio che si chiude in tre mesi, dando certezze e risparmiando costi? Mi sembra che in una visione veramente democratica l'arbitrato lo sia, in una prospettiva tipicamente occidentale, molto di più e molto meglio che non il vecchio processo, questo sì classista ed incupito nella sua burocraticità ed opacità.

a ribadire semplicemente tre punti. Con questo provvedimento, una volta approvato, verrà rafforzato il criterio di trasparenza della pubblica amministrazione, del *benchmarking* comparativo tra pubbliche amministrazioni; con esso vengono resi omogenei gli ordinamenti dei vari comparti e, soltanto per fare un esempio, viene valorizzato l'apporto e il ruolo del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.

nel sistema delle relazioni anche industriali e di lavoro all'interno della pubblica amministrazione.

cito, da ultimo, il collega Pichetto Fratin, che ha sottolineato la necessità di affrontare riforme strutturali in materia di ammortizzatori e di mercato del lavoro. Quelle riforme di carattere generale e sostanziale cui ci riferiamo

il collega Castro di avere la compiacenza di non prendersi gioco dell'opposizione riducendo a macchietta le valutazioni che l'opposizione propone,

assolutamente parziali; certo, alcuni di questi connotati hanno un profilo riformatore, ma assolutamente insufficiente rispetto al perimetro ed alla gravità dei problemi che dobbiamo affrontare. Non voglio fare del "benaltrismo", ma

anche qualora condivisibili, sono comunque assolutamente parziali e non commisurate all'entità dei problemi. Infine, sulla necessità di mantenere la coesione sociale e sul ruolo che rispetto a questo obiettivo avrebbe la riforma del contenzioso e la proposta che ci viene dalla maggioranza in materia di arbitrato, il collega Castro ha sottolineato ripetutamente che la proposta della maggioranza valorizza la possibilità del confronto e dell'accordo fra le parti negozialmente concordati. Abbiamo fortissimi dubbi che questo possa avvenire; siamo certi, anzi, del contrario. Se ci sbagliamo invitiamo il collega Castro e la maggioranza ad accogliere la nostra proposta che limita all'ambito negoziale fra le parti l'esercizio dell'arbitrato e lo svolgimento del medesimo. Vedremo,

diritti dei lavoratori e quelli delle imprese, che devono guardare il proprio futuro in un contesto di modernizzazione, che fornisca loro strumenti per

Presidente, mi rivolgo in particolare ai relatori, alle loro repliche ed al Governo. Nonostante le argomentazioni molto forbite e convincenti del senatore Castro, almeno per quanto mi riguarda credo fatte in perfetta buona fede e non soltanto perché è relatore di maggioranza,

Davvero non ne vedo la ragione; davvero non mi sembra sia questa una risposta alla crisi. Sono d'accordo - e l'abbiamo detto, quindi è inutile dire che noi non siamo d'accordo - sulla semplificazione, su alcune norme, sull'aspettativa, dove abbiamo pure espresso alcuni pareri.

e siamo d'accordo, che d'ora in poi i *part-time* si chiedono e si ottengono anche con una valutazione dell'amministrazione; questo mi sembra giusto. Ma voler ritornare su un *part-time* già ottenuto mi sembra penalizzante, inutile e dannoso.

metterli dentro al comitato del *mobbing* (che è paritetico, perché previsto dal contratto), stravolgere per questa via anche il *mobbing*, che aveva una sua specificità (perché il contratto lo prevedeva)

Signora Presidente, intervengo a questo punto del dibattito - fermo restando che il confronto parlamentare sarà arricchito dalla pluralità degli emendamenti e dal confronto sugli emendamenti stessi

relatori, del Presidente della Commissione e dei senatori di maggioranza hanno illustrato ampiamente il senso, il significato, l'importanza e il rilievo del disegno di legge che stiamo affrontando, pur trattandosi di un provvedimento che, per diverse ragioni e per diverse motivazioni, ha un carattere che non sempre è facile da condurre ad armonicità degli interventi e degli argomenti. subisce una sorta di difetto di sistema, che presumibilmente sarà definitivamente superato con la nuova idea che è emersa in maniera unanime

Credo tuttavia che il contributo dell'opposizione nel corso di questi mesi sia stato utile, importante e significativo. Non vorrei che dimenticassimo il lavoro che è stato svolto in Commissione.

per cercare di affrontare alcuni nodi in maniera equilibrata. Non so se siamo riusciti a trovare il punto di sintesi rispetto ad alcune questioni fondamentali. ad esempio, all'arbitrato. Ricordo a me stesso che una delle questioni maggiormente dibattute in Commissione è stata quella di trovare un punto di equilibrio che, nel contempo, determinasse un recupero di efficacia, di efficienza, di semplificazione e di rapidità, senza però pregiudicare il sostegno e la partecipazione nel processo della decisione delle parti sociali e, quindi, il ruolo e la funzione, in particolare delle parti sociali, rispetto alle modificazioni che intervengono. Lo dico anche in relazione all'intervento

è stato esattamente quello di evitare che l'arbitrato si riducesse ad un rischio di eccessivo individualismo, (diciamola così per intenderci); la ricerca è stata volta a trovare un punto di equilibrio, che a mio avviso è stato trovato. Poi, per il resto, lei ha ragione, senatore Pardi: è vero che siamo in presenza di una condizione che potremmo definire di solitudine dell'inoccupato, del disoccupato, del lavoratore che perde il posto, ma essa non è a mio avviso attribuibile alla vecchia concezione del rapporto di forza e di debolezza tra le parti, quasi con una sorta di rovesciamento dell'identità collettiva che presiedeva una volta e che invece oggi si è trasferita sul versante dell'impresa. Mi sembra che non sia questa la dimensione, il problema, l'impostazione, l'approccio culturale. C'è il tema della solitudine, e rispetto ad esso non c'è solo la risposta dei dei soggetti che si auto-organizzano nell'associazione, nel sindacato e in quant'altro, ma c'è lo sforzo per garantire i servizi e per determinare punti di riferimento in cui quella solitudine

Sappiamo bene che tali problemi sono di fronte a noi e che non è questo il provvedimento capace di risolvere questi aspetti del mercato del lavoro che non funzionano ancora. Anche in anziché salutare come elemento significativo la presenza di più attori nell'incrocio offerta‑domanda, molte volte ci soffermiamo ancora su questa sorta di monopolio statale dell'incrocio offerta-domanda come se la funzione pubblica non potesse essere svolta da altri soggetti, come se le università, i consulenti del lavoro e tanti altri soggetti del privato sociale non dovessero essere chiamati a questo sforzo per dare una risposta di pluralità

che il tempo delle riforme strutturali ancora non è arrivato perché, all'interno di una crisi i cui connotati non sono ancora del tutto precisi, delineati e dimensionati, è il caso di attendere l'assestamento

un primo passo verso la costruzione, finalmente, di un sistema organico di riforma delle tutele e degli ammortizzatori sociali. Non voglio entrare nel merito

nel 2001, quando vi era la delega aperta del Governo D'Alema che pretendeva di fare la riforma degli ammortizzatori sociali a costo zero. Avvertiamo tutti l'esigenza di recuperare il massimo di corresponsabilità possibile rispetto a scelte strutturali che non sono state fatte e che non possono essere utilizzate come arma di contestazione o di propaganda di schieramento. Infatti, esse attengono ad una difficoltà di sistema che si è manifestata sia sul versante

e non alla dimensione macro, come era nel modello di carattere fordista della grande fabbrica. Sicuramente il provvedimento al nostro esame non affronta in maniera determinata e strutturale alcuni argomenti, ma segnala

parere non ostativo». «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sul testo a condizione che, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'articolo 2-*bis* le parole: "articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549" siano sostituite dalle seguenti: "articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502". Esprime inoltre parere di semplice contrarietà sugli articoli 27-*undecies* e 27-*sexiesdecies*. Per quanto riguarda gli emendamenti, esaminate le proposte fino all'articolo 27, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.201, 4-*bis*.304 (testo 2), 7.0.11, 8.200, 14.0.200, 22.200, 27-*sexies*.200, 27-*decies*.200 e 27-*undecies*.200. Esprime poi parere di semplice contrarietà sulle proposte 1.200, 6-*septies*.201 e 14.300. Esprime inoltre parere di nulla osta su tutti i restanti emendamenti ad eccezione della proposta 14.0.201, sulla quale il parere è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, a che al comma 5 la parola: "valutato" sia sostituita dalla seguente: "determinato" e le parole: "5 milioni", ovunque ricorrano, siano sostituite dalle seguenti: "10 milioni". Il parere è rinviato sugli emendamenti riferiti a partire dall'articolo 28».

commi 2-*ter* e 2-*quater*, del Regolamento, sono inammissibili, per estraneità all'oggetto del disegno di legge collegato in esame, i seguenti articoli introdotti nel testo nel corso della trattazione in Commissione, in quanto non riferibili alla materia del lavoro pubblico e privato: - 2-*quater* (Disposizioni per

a lungo esaminata e sostenuta anche da parte della maggioranza; quindi, mi aspetterei un'attenzione, in particolare dai colleghi della Lega. Per quanto riguarda l'emendamento 1.200, riteniamo che la materia venga regolata

si chiede di sopprimere il comma 1-*bis* perché il diritto al pensionamento anticipato per chi svolge lavori usuranti non è determinato dai requisiti necessari

Più avanti ancora si dice addirittura che questo diritto fondamentale per chi svolge lavori pesanti e particolarmente usuranti deve essere legato al numero delle pratiche che verranno accolte. Penso che una cosa del genere non si sia mai vista, vale a dire condizionare, legare al pensionamento anticipato per chi svolge lavori così pesanti alle disponibilità del bilancio o addirittura all'accettazione delle domande. Guarda caso, quando sono in discussione

parere conforme al relatore.

nel testo dell'articolo proprio il tema dell'individuazione del rapporto di strumentalità tra INAIL ed ISPESL. Chiediamo pertanto di comprendere meglio la *ratio*

dal senatore Vizzini prevede la doverosità dell'intervento di primazia organizzativa dell'INAIL sull'ISPESL, limitandosi ad affermare che non vi è tuttavia una subordinazione strutturale, come ente strumentale, dell'ISPESL nei non vi è una trasformazione della struttura organizzativa, bensì il riconoscimento della primazia funzionale dell'INAIL sull'ISPESL, nella mera necessità di garanzia del coordinamento sulle attività a presidio della sicurezza sui luoghi di lavoro.

di un articolo che è stato modificato e migliorato a seguito del dibattito avvenuto in Commissione, con un apporto significativo anche del nostro Gruppo. Rimangono però, a nostro modo di vedere,

è consapevole della necessità di razionalizzare e di fare un po' di ordine presso questi enti vigilati. Ci rendiamo infatti conto della sovrapposizione di competenze,

Non da ultimo vi è il tema del personale. Pensiamo che vadano salvaguardate le risorse umane all'interno di questi enti attraverso processi di mobilità.

della Commissione sugli infortuni sul lavoro. Qui parliamo dell'ISPESL e dell'INAIL, cioè degli enti che sono preposti a

Signora Presidente, l'articolo 4, di cui con il presente emendamento chiediamo la soppressione, modifica la disciplina relativa alle sanzioni amministrative e civili previste per il caso di impiego di personale non risultante dalle scritture o dai documenti obbligatori. In particolare, con l'articolo 4 si introduce una sanzione amministrativa più lieve per coloro che, pur avendo utilizzato lavoro irregolare, abbiano successivamente regolarizzato lo stesso lavoratore e si modifica la disciplina relativa all'entità delle sanzioni civili per l'utilizzazione di lavoro sommerso. inoltre dall'applicazione delle sanzioni amministrative relative all'impiego di lavoro sommerso coloro che non abbiano dolosamente occultato il rapporto di lavoro. Si osserva che tale articolo nasconde in realtà la volontà del legislatore di impedire la corretta applicazione delle discipline varate dal precedente Governo al fine di far emergere il lavoro nero e garantire così la sicurezza nei luoghi di lavoro.

in realtà il solito emendamento, che periodicamente riproponiamo, che riguarda il grave sfruttamento del lavoro. In proposito abbiamo presentato anche un disegno di legge che non è mai stato messo all'ordine del giorno dei lavori della Commissione, ma che comunque tocca un problema essenziale, che è quello appunto del grave sfruttamento del lavoro dei cittadini sia italiani sia stranieri. Naturalmente, tutto questo crea non solo un danno per l'economia e uno sfruttamento del lavoro, ma anche una conflittualità riguardo al fatto che vi sono imprese che si reggono

si parla soltanto di un'integrazione di dati e non già di un ritardo in una comunicazione.

in diverse occasioni e in interviste su vari giornali, ha preannunciato un aumento dei contributi previdenziali per per tutta l'area del lavoro parasubordinato, cioè delle collaborazioni autonome continuative. Su questo terreno ricordato che esistono collaboratori autonomi continuativi sostanzialmente equiparabili ai lavoratori subordinati, ma esistono anche collaboratori autonomi che sono sostanzialmente dei liberi professionisti, per i quali il contributo grava sul fatturato al lordo delle spese di produzione del reddito.

in questi casi di vero lavoro autonomo, una contribuzione che supera il 50 per cento dell'utile del lavoratore. Credo che sia essenziale ed urgente che il Parlamento affronti questo problema, per arrivare alla indispensabile

Altrimenti, noi perpetuiamo una sostanziale rapina ai danni di una categoria importante, che supera il milione e mezzo di lavoratori realmente autonomi iscritti alla gestione separata dell'INPS.

vorrei iniziare con la lettura di una frase, per far capire il problema di cui voglio parlare: «La miseria non sia zittita, ma piuttosto ascoltata per essere superata. A vincere deve essere sempre l'infinita dignità dell'essere umano. Chi ha alte responsabilità deve ascoltare l'invocazione che viene da tante forme di miseria, di ingiustizia e di solitudine». È una frase del cardinale Dionigi Tettamanzi, arcivescovo di Milano (la diocesi più grande del mondo). Egli ha usato queste parole l'altro giorno, quando è stato sgombrato il campo rom di via Rubattino. Nessuno vuole che la popolazione rom e nomade viva in campi non adeguati, essere sgombrato solo quando le istituzioni pubbliche sono in grado di dare una risposta positiva ed alternativa a quella forma di miseria, perché quella è sicuramente una forma di miseria. Non siamo qui a difendere i campi rom.